Grazie,

di dare dei suggerimenti per migliorare la lotta alla criminalità organizzata, che non può essere fatta, evidentemente, solo catturando i latitanti, ma anche, e soprattutto, riappropriandosi del controllo del territorio - ciò che sta a cuore specie a chi si occupa di questa materia (mi riferisco alle procure distrettuali) - dando la possibilità di utilizzare le

abbia dato conto di quella che è stata l'attività della Commissione su questo provvedimento, che ha portato ad un'unanimità di posizioni. Una posizione, ripeto, ben illustrata dal relatore e che ha trovato espressione nell'intervento del senatore Li Gotti, che ha già indicato l'intenzione di ritirare tutti gli emendamenti da lui presentati, in quello spirito di collaborazione che ha caratterizzato l'attività

L'articolo 2 del disegno di legge sicurezza ha trovato l'unanimità del voto sia alla Camera che al Senato

Parlamento. La concretizzazione della lotta alla mafia non è fatta di parole, di un mero vantarsi di alcune iniziative legislative. vantare il fatto che questo provvedimento ha visto una serie di emendamenti del Governo; ma non è questo lo spirito che anima il Governo nella valutazione complessiva dell'azione che che tutto lo Stato deve condurre. Ho già detto in un'altra seduta di avere delle critiche tecnico-giuridiche, delle perplessità, perplessità è però di ordine politico, perché il reato di concorso esterno in associazione mafiosa determina da parte dei cittadini la percezione di un qualcosa che normalmente è tollerato e che in quel determinato processo diventa invece reato. La vera rivoluzione che era quella che ci insegnavano Rocco Chinnici e Giovanni Falcone, di cui ero amico e con i quali ho lavorato nella lotta alla mafia (una lotta che non è fatta di parole, senatore Lumia, o di rivendicazioni, che non portano

essa è il frutto dell'azione complessiva che c'è stata tra Governo e Parlamento e che ha fatto percepire agli uomini delle forze dell'ordine e alla magistratura che vi era una solidarietà complessiva dell'intera classe politica?

che invece rifiuto. Ripeto che voglio rivendicare quanto il Governo ha fatto, perché solo nella collaborazione

possibilità di quel tipo, furono organizzate riunioni con tutti i procuratori generali d'Italia, il Ministro dell'interno, che era l'onorevole Cossiga, e il Ministro della giustizia, della giustizia, per creare quel raccordo e quella circolarità di notizie tra le procure generali, che ancora non esisteva, perché non c'era ancora un sistema di coordinamento. È questa la logica che ci deve ispirare nell'esaminare questo e altri provvedimenti del

poiché non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti presentati, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

senatore Balboni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Conseguentemente appare assolutamente logico e necessario far sì che anche la competenza

funzionale, civile e sociale delle attribuzioni territoriali e demografiche degli uffici giudiziari. Nel caso specifico, il mio personale pensiero, e anche quello di molti altri colleghi del mio Gruppo,

o in via generale o per casi specifici, alla redistribuzione delle circoscrizioni giudiziarie, ciò deve essere ispirato ad un principio prioritario e fondamentale, quale quello del riequilibrio demografico e territoriale. A modello di quanto si è cominciato a fare per alcuni tribunali di città metropolitane e per i loro tribunali finitimi, il principio deve essere non quello di sopprimere i cosiddetti uffici giudiziari minori, che è un gravissimo errore dal punto di vista sociale, economico, istituzionale e anche sotto il profilo dell'amministrazione della giustizia nell'interesse dei cittadini, ma quello di riequilibrare le competenze territoriali e demografiche. è semmai necessario scorporare parte delle competenze demografiche e territoriali dai tribunali troppo grandi e troppo congestionati per accorparle a tribunali finitimi più piccoli o addirittura considerati (sia (sia pure con opinabili parametri) sottodimensionati. Quindi, ove si dovesse mettere mano alle circoscrizioni giudiziarie, in generale o per casi specifici, deve essere prioritariamente uno: né quello della soppressione, né quello degli accorpamenti, né quello degli accentramenti, bensì quello del riequilibrio territoriale.

per vedere se siano ben distribuite le competenze, se sia equilibrato il carico della popolazione, del territorio e quindi anche del lavoro, della competenza civile e penale. Nessuno impedirebbe che questo principio, che ho ribadito come prioritario per i tribunali, possa e debba valere anche per le corti d'appello: per le corti d'appello: quelle troppo cariche e troppo grandi potrebbero essere sgravate mediante distacco di porzioni della popolazione e del territorio, per accorparle a corti d'appello finitime, confinanti. Alcuni altri propongono, alle volte oggettivamente e alle volte per spinte locali, di istituire nuove corti d'appello, cadendo in una singolare contraddizione che in maniera un po' divertita ho più volte colto: colto: mentre reclamano a gran voce la soppressione di tribunali o di uffici decentrati, che presidiano il territorio e servono le comunità locali, poi chiedono l'istituzione di nuove corti d'appello. È evidente il particolarismo e l'unidimensionalità di questa impostazione.

due ragioni. Innanzitutto, l'incidenza territoriale e demografica sull'equilibrio del lavoro e della funzionalità dei due uffici giudiziari (quello che perde territorio e quello che lo acquista) non è stravolgente (tuttavia, non vi sfuggirà che all'articolo 3 del testo del disegno di legge pur si prevede che con decreto del Ministro della giustizia debbano essere apportate opportune modifiche alle piante organiche: quindi, una qualche modificazione in realtà si induce). corrisponde ad esigenze orografiche, territoriali, civili, economiche e perfino, *lato sensu*, culturali, che hanno legittimato non solo il trasferimento della competenza amministrativa da una Regione all'altra, ma che nel caso specifico, per l'efficienza e la razionalità del servizio giudiziario, giustificano anche il trasferimento di competenza Ho voluto sottolineare, cogliendo l'occasione di questo provvedimento che in sostanza è largamente condiviso, che anche nella redistribuzione e nel trasferimento di competenze territoriali e demografiche sul piano giudiziario si deve sempre guardare all'aspetto dell'omogeneità e della gravitazione economica, sociale e alla consistenza orografica dei territori, oltre che ai collegamenti,

vi è un adagiarsi su certe forme di apparente comodità di aggregazione territoriale, che però non corrisponderebbero, nel caso specifico, alla razionalità della redistribuzione delle competenze in termini giudiziari. infatti, essere obiettivo principale dell'amministrazione della giustizia il rendere efficiente il proprio servizio in collegamento con i territori e, quindi, redistribuire equamente equamente ed equilibratamente tali competenze. Per queste ragioni che, come vedete, sono state criticamente esaminate e valutate, siamo sicuramente orientati, insieme ai firmatari del disegno di legge, a votare a favore dello stesso.

questo provvedimento, in larga parte condiviso, salvo per un aspetto che poi il collega Morri esporrà in riferimento al Comune di Montecopiolo, quanto piuttosto intervenire per ricordare all'Aula e al collega Benedetti Valentini

una difficoltà degli uffici giudiziari sotto il profilo degli strumenti e degli apporti dei funzionari dell'amministrazione della giustizia, ossia i cancellieri e segretari, i quali sono stati ridotti nel numero in rapporto a piante organiche sottodimensionate, e in relazione ad un difetto ormai palese della volontà

La riforma delle circoscrizioni giudiziarie diventa quindi qualcosa di indispensabile per la razionalizzazione delle risorse. Noi non possiamo accettare un discorso che parta da una posizione preconcetta nei confronti di una riforma che viene sollecitata da tutti gli operatori della giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura nella precedente legislatura ha concluso la propria operatività con una proposta sulla riforma delle circoscrizioni giudiziarie; gli avvocati, nelle varie composizioni associative, richiedono un diverso accorpamento degli uffici giudiziari per rendere più efficace la giustizia; la magistratura associata denuncia costantemente

Se non si procede ad una riforma delle circoscrizioni giudiziarie e ad una razionalizzazione delle stesse, mancheranno sempre mezzi, strumenti, operatori, magistrati. Poiché si deve lavorare sull'esistente,

«La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione, per il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime per quanto di competenza parere non ostativo». parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "sono apportate" siano aggiunte le altre: ", nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,". Esprime poi parere non ostativo sugli emendamenti ad eccezione della proposta 3.0.100 sulla quale il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale».

è stato inserito, insieme a sette Comuni della zona del Montefeltro che hanno compiuto tutto l'*iter* per il passaggio dalla Regione Marche all'Emilia-Romagna, un Comune che invece rimane a tutt'oggi nel territorio della Regione Marche. Si tratta di un piccolo Comune che porta il nome di Montecopiolo.

che è più vicino, così come già oggi avviene per i Comuni contermini a questo, come quello di Carpegna e altri confinanti. In caso

ripeto, è nel mandamento del giudice di pace di Novafeltria. Una sentenza del giudice di pace di Novafeltria, per effetto della legge che noi oggi approviamo, potrà essere impugnata soltanto davanti al tribunale di Rimini. Se noi non mettessimo Montecopiolo insieme agli altri Comuni, che fanno tutti parte del mandamento del giudice di pace

la Commissione giustizia ha deciso di inserire Montecopiolo tra i Comuni oggetto del presente disegno di legge. Data la brevità, do lettura all'attenzione del senatore Filippo Berselli: «Il sottoscritto Alfonso Lattanzi, sindaco di Montecopiolo, a nome di tutta la cittadinanza, chiede che venga approvato il passaggio del Comune di Montecopiolo al circondario

quindi una richiesta esplicita, e non vedo, in ragione di queste motivazioni tecniche, perché non si debba accedere ai desideri, legittimi e giustificati, del Comune di Montecopiolo.

infatti far presente ai presentatori dell'emendamento 1.100, di cui chiedo il ritiro, che non è la prima volta

c'è un gruppo di Comuni che sono aggregati al Comune di Cassino, quindi al Lazio, esclusivamente perché

risolta, come ricordato dalla senatrice Della Monica, con una revisione delle circoscrizioni che non può essere operata togliendo un solo Comune a quello che era il vecchio mandamento, ciò che altererebbe quelle che sono le competenze in base all'attuale disciplina.

di una prova seduta stante della pertinenza di quelle poche e modeste considerazioni che mi sono permesso di fare in discussione generale, mi è mi è stata ora offerta su un piatto d'argento. Ho detto prima che è sbagliato, da un punto di vista generale, concettuale e funzionale, rendere l'attribuzione di competenza territoriale legata a quella di carattere amministrativo e che, anzi, dovremmo, non dico scordarcela del tutto, ma quasi. Ancor meglio, il fatto che un sindaco, o persino un Consiglio comunale, si pronuncino in una certa direzione in materia giudiziaria, naturalmente di importante rilievo democratico, non è decisivo ai fini dell'assunzione delle nostre responsabilità politiche e legislative, se non vogliamo essere pigri o demagogici, da questo punto di vista. Quando si mettono le mani sulle circoscrizioni giudiziarie, lo so che ci sono i mandamenti dei giudici di pace che in qualche modo si rifanno a quelli delle procure,

di quasi tutta l'Italia) nei quali sarebbe persino opportuno scorporare comuni e territori comunali da certi mandamenti di competenza dei giudici di pace perché rientrino in questa redistribuzione territoriale. Nel caso specifico, vi debbo dire che mi trovo in serissimo imbarazzo, perché

giudiziarie, sia per quanto riguarda i circondari dei tribunali, *et ergo* della corte d'appello, sia per quanto attiene al mandamento del giudice di pace, provvedendo a sistemare in maniera sintonica le due questioni. Potrebbero invece prevalere

le parole suggerite da quella Commissione per garantire che non vi saranno ulteriori nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Colgo l'occasione, visto che ho la parola, per annunciare che, alla luce dell'inserimento del Comune di Montecopiolo fra i Comuni che vengono trasferiti alla competenza del tribunale di Rimini e della corte d'appello di Bologna, credo sia necessario cambiare il titolo della legge,

l'utilizzazione ottimale delle risorse. In una parola, l'organizzazione. Governo dovrà dare atto che mentre si producono o si annunciano provvedimenti in tema di giustizia, in tema di organizzazione e miglioramento della macchina giustizia lo stesso è totalmente assente,

Quello della geografia giudiziaria è un problema antichissimo: risale a un secolo e mezzo fa. Si dice che per poter mettere mano alla geografia giudiziaria servano le legislature lunghe, quanto ovviamente mettere mano alla geografia giudiziaria significa provocare le cosiddette guerre di campanile, sicché chi decide di fare l'opera meritoria dovrà poi ammortizzare i contraccolpi della stessa. Ma è un problema che esiste.

ad esempio degli uffici dei giudici di pace. Ci sono uffici che hanno iscrizioni in numero di dieci cause in un anno, e non si riescono a chiudere. Siamo riusciti a farlo esclusivamente per Cortina d'Ampezzo, sede del giudice di pace, che chiese che venisse chiuso l'ufficio perché non lo voleva. l'unico intervento che si riuscì a fare; per il resto non si riesce, in quanto il territorio rivendica il prestigio di avere un ufficio giudiziario. Conosco anche le battaglie, in gran parte da me condivise, portate avanti dal senatore Benedetti Valentini con l'associazione dei piccoli tribunali. È vero, esiste la realtà dei piccoli tribunali, e noi dobbiamo tutelare alcune realtà ormai storicamente consolidate con la presenza degli uffici giudiziari: ma la razionalizzazione è necessaria. Pensate che in Calabria esistono due corti d'appello con poco più di due milioni di abitanti; nel Lazio, con oltre cinque milioni di abitanti, c'è una sola corte d'appello. Questo significa che esiste un problema di organizzazione. In Puglia c'è una corte d'appello con un unico tribunale, la corte d'appello di Taranto (unico tribunale, Taranto); poi abbiamo la corte d'appello di Lecce e la corte d'appello di Bari. Nel Veneto c'è una sola corte d'appello. Vi è una serie di problemi che devono essere affrontati.

Il Ministro della giustizia nel 2010 ha annunziato che della riforma della geografia giudiziaria neanche se ne parla;

Ma la politica deve farsi carico di tale questione. Non risolveremo i problemi della giustizia se non affrontiamo questa riforma

Annunciamo che vogliamo fare i processi brevi con una macchina non funzionante. Dobbiamo prima aggiustare la macchina, e poi possiamo fare i processi brevi, perché diventeranno tali come conseguenza di una macchina aggiustata. Sulla macchina, invece, il Governo non intende intervenire. Questa è la più grave contraddizione che dimostra la strumentalità degli annunci della riforma della giustizia: non è una riforma, sono esclusivamente espedienti *ad usum Delphini.

credo che su questo provvedimento ci sia il consenso di tutta l'Assemblea, per ovvie ragioni. Innanzitutto, rispetto al *referendum* che si è svolto il 17 ed il 18 dicembre 2006,

Quindi, mediante il disposto della legge n. 117 del 3 agosto 2009, il distacco di questi sette Comuni è stato avviato. Ma tutto questo risponde, come già diceva il senatore Benedetti Valentini, ad una esigenza di tipo culturale, antropologico, orografico di un territorio che è quello dell'Alta Valmarecchia, che necessita di essere aggregato alla realtà del Comune di Rimini e quindi dell'Emilia-Romagna. Il problema, così come è stato evidenziato anche da altri interventi, è quello della ridefinizione delle circoscrizioni. Ma, se noi continuiamo comunque ad affrontarlo per piccoli *spot*, credo che non facciamo un buon servizio alla causa, ancorché, per quello che riguarda il provvedimento di cui discutiamo, è fatto di necessità, per cui, ovviamente, il legislatore deve operare in conseguenza a quanto è avvenuto ed è stato disposto mediante *referendum*, con l'accettazione di quello che veniva dal *referendum* stesso. dal *referendum* stesso. La questione della ridefinizione delle circoscrizioni, che attiene ad un più ampio riordino di tutto il comparto giustizia per il suo migliore funzionamento, non deve prevedere semplicemente un tema un tema quale quello della razionalizzazione, che troppo spesso viene concepito e definito in maniera molto ragionieristica con tagli che non incidono sulla qualità del servizio, quando il servizio giustizia è uno dei più qualificanti di un Paese democratico. Quindi, credo che alla parola razionalizzazione vada comunque abbinata anche un'altra parolina significativa. La razionalizzazione richiede non solo, a volte, dei tagli, e quindi una normalizzazione delle realtà, ma anche, e soprattutto, una implementazione di risorse, al contempo umane, tecnologiche e finanziarie. Una razionalizzazione che valga la pena fare richiede soprattutto questo: non soltanto lo spostamento

appunto, si dice che «entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Pesaro e di Rimini».

difficoltà le realtà locali che stanno già lavorando a tal fine. Queste ultime non si vedono tolti i provvedimenti: vengono lasciati lì. Quindi, con minore personale, non so come potrebbe andare a finire.

con una considerazione. Naturalmente abbiamo constatato, anche dal dibattito di questa mattina, quanto sia interessante, e anche obbligato, mettere mano al tema della riorganizzazione delle circoscrizioni, registriamo, anche in questo piccolo saggio introduttivo - così io lo considero - i tanti punti di vista che ci sono Vorrei accompagnare questa riflessione con un giudizio del Partito Democratico, che è aperto alle soluzioni che portano ad una maggiore efficienza dell'ordinamento giudiziario, ritenendo che l'approccio debba essere quello di partire dalla tutela dell'utenza, perché la soppressione o la riorganizzazione di una circoscrizione è tema che riguarda non solo gli operatori giudiziari ma soprattutto l'utenza. Quindi, annunciamo voto favorevole al provvedimento

ho ascoltato con attenzione l'intervento del senatore Li Gotti, che ha affrontato il tema dell'esigenza di rivedere le circoscrizioni giudiziarie. È un tema certamente all'ordine del giorno di chi si interessa di giustizia: sappiamo che ci sono Regioni, come l'Emilia-Romagna, dove vi è un tribunale in ogni capoluogo di provincia e non di più, e dove vi è una sola corte d'appello, il cui distretto coincide appunto con la medesima Regione. Anche noi siamo sensibili alle esigenze dei piccoli Comuni, e quindi, a maggior ragione dei piccoli tribunali; però, sappiamo anche che vi sono Regioni in cui, anche per retaggio storico, vi sono tanti piccoli tribunali. Voglio ricordare al senatore Li Gotti e ai tanti colleghi dell'attuale opposizione che contestano il ministro

e dal 2006 al 2008, le circoscrizioni giudiziarie non sono state riviste nel nostro Paese. È vero quanto dice il senatore Li Gotti: è materia estremamente delicata, come è delicata la materia della soppressione di determinate Province. Tutti noi saremmo d'accordo per ridurre il numero delle Province; però, quando andiamo a porre mano a questo tema, ci scontriamo con esigenze di carattere territoriale e localistico. Lo stesso discorso si può fare per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie,

che sono molto più vicini a Rimini di quanto non lo siano a Pesaro e che, per transitare verso Pesaro, debbono passare per Rimini:

le cui vie di accesso per Pesaro passano attraverso la città di Rimini. Vi posso dire che questo Parlamento, con un voto pressoché unanime, approvò una legge che trasferiva dal punto di vista amministrativo quei sette Comuni dalla Provincia di Pesaro e Urbino alla Provincia di Rimini. È stato giustamente ricordato dalla senatrice Sbarbati che ciò avvenne previo *referendum,* che si concluse con un risultato pressoché plebiscitario a favore delle attese e delle esigenze di quelle popolazioni.

Riteniamo che questo disegno di legge debba essere approvato, non solo perché - ripeto - condiviso dal Senato della Repubblica, ma soprattutto perché va incontro alle aspettative delle popolazioni

opportuno fare una precisazione, proprio per evitare dei fraintendimenti, quali quelli che si sono verificati questa mattina anche con il rappresentante del Governo. La precisazione riguarda proprio l'espressione del parere della 5a Commissione. 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dico questo, perché, in seno alla 5a Commissione, anche il rappresentante del Governo aveva espresso delle perplessità in ordine all'articolo 6 che concerne la clausola

della 5a Commissione, ma soprattutto per invitare il Governo, in una materia così importante come la lotta alla criminalità a livello internazionale,

Presidente, colleghe e colleghi, insieme al senatore Asciutti abbiamo vergato la relazione allegata

approvato già dalla Camera dei deputati e lungamente dibattuto nella 7a Commissione del Senato, riguarda la nuova disciplina del prezzo dei libri. È un disegno di legge - mi permetto di sottolinearlo, signora Presidente, colleghe e colleghi - meritevole di attenzione e di cura. cura. Il tema del prezzo del libro, infatti, lungi dall'essere una questione meramente economica, attiene da vicino alla salvaguardia della cultura nelle sue forme più ampie. Vale a dire, il prezzo assume un ruolo persino superiore al suo stesso oggetto, ed è quasi una metafora del tema generale della lettura. Del resto, il diavolo si nasconde spesso nei particolari. del centenario della nascita di Mc Luhan, e alla vigilia di una importantissima Fiera del libro a Torino, dobbiamo considerare finalmente il libro la parte profonda del nostro cervello. La lettura rappresenta l'unico modo per trasformare il linguaggio in pensiero ed il libro - ecco il tema - non è un *medium* tra gli altri o come gli altri: è, in un certo senso, l'identità medesima della conoscenza. Non morirà mai, neppure nell'era di Internet e della Rete. Senza libri verrebbe meno l'essenza stessa dell'umanità. Ecco perché parlare del libro, ancorché assunto da una specifica finestra, quella del prezzo - ci arriveremo tra poco vuol dire segnalare il grado di civiltà dell'Italia nel villaggio globale. Il libro è l'io conoscente, che si reifica in quella tavoletta - il nostro angolo visuale - che ha accompagnato le diverse stagioni della comunicazione. Intitolata in diverse maniere, la radice etimologica della parola libro è legata proprio all'oggetto fisico, il supporto per la scrittura. Dopo le lunghe stagioni delle culture orali, ecco il libro, che diventa il modo di essere del nostro pensiero. L'UNESCO suggerisce una definizione di libro quale «pubblicazione a stampa, non periodica, di almeno 49 pagine», nella quale compaiono elementi esterni rispetto alla pura considerazione del supporto, come i concetti di pubblicazione e periodicità.

Il libro rimane libro anche nella stagione del grande mutamento tecnologico. Non è quindi una struttura fisica; è un concetto più profondo: la coscienza intellettuale. Così anche la libreria, che è il sottotesto di questo testo che vogliamo valorizzare, è in un certo senso il tempio laico dei saperi. Attorno alla nuova biblioteca digitale si gioca - come sapete, Presidente, colleghi e colleghe, è in atto un dibattito internazionale - la più colossale guerra simbolica del nostro tempo, ivi compreso il nuovo concetto di proprietà intellettuale, o *copyright*. I libri sono un bene comune. Non appartengono alla versione «mercatista» del mercato, da leggere - questo ultimo - con occhiali molto diversi quando si parla di un bene particolare come la lettura. Ecco perché sentiamo l'esigenza, come è stato nel passaggio alla Camera nel testo che ha come primo firmatario il collega Levi, di legiferare anche sul prezzo del libro. Non solo, è una sequenza di una riforma più ampia, cui davvero con spirito unitario rinviamo per una più compiuta iniziativa attorno al tema così cruciale dei nostri saperi. Il futuro si gioca anche qui, e se il libro ci sarà saremo meno colonia televisiva e più luogo emancipato, perché i libri sono plurali: c'è una varietà che l'omologazione del tubo catodico, ora digitale, non ci assicura. Nell'era dei tagli alla, nella e della cultura, guai alla morte in diretta delle case editrici di minori dimensioni o delle librerie non legate ai maggiori gruppi! Sarebbe la fine: non già del libro vecchio stile, sussunto da quello *on line* ma, al contrario, sarebbe il falò, come in Fahrenheit dei messaggi e dei contenuti, essenziali per qualsiasi processo tecnologico. I contenuti digitali non sono meno importanti, anzi, forse più ancora di quelli dell'altra stagione.

degli incunaboli, ma lo è nell'epoca dei «*Wreader*», i nativi digitali che sono insieme lettori e scrittori, nella Rete, della Rete. Gutenberg, Marx e tanti autori ci hanno ammonito sull'innovazione tecnologica e il suo valore, così come tanti studiosi - riassumo velocemente - ci hanno però spiegato - da Bolter e Grusin, sulla "rimediazione", a Fidler, sulla trasformazione e la "mediamorfosi" dei mezzi di comunicazione - che il libro non muore, si trasforma, e si rimedia con l'innovazione tecnologica. La sua essenza rimane ancora più significativa, tant'è vero che, in un recente volume, molto gradevole, Jean Claude Carrière e Umberto Eco ci hanno detto: «Non sperate di liberarvi dei libri. Il libro si appresta a fare la sua rivoluzione tecnologica, ma ci troviamo di fronte - aggiungono - a uno strumento che per quante mutazioni abbia subito» - e per quante ne subirà, aggiungiamo noi «si è comunque mostrato di una straordinaria fedeltà a se stesso. Il libro appare a tutti noi una sorta di "ruota del sapere e dell'immaginario" che le rivoluzioni tecnologiche annunciate o temute non elimineranno». Venendo

dei guai in vista. John Makinson, amministratore delegato della Penguin, che nel corso della conferenza di presentazione dei nuovi titoli per iPad, utilizzò - anzi, si lasciò sfuggire - il termine «consumatori» invece di «lettori».

quantitativi - con Grecia e Portogallo un triste primato europeo: il più basso indice di consumi culturali. Dai musei ai teatri, dai giornali e libri, molti degli italiani - stregati dalla televisione o dal cellulare

la spesa per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche pubbliche, altro punto dolente, è scesa dai 65,5 milioni di euro del 2005 ai 48 milioni di euro del 2008;

lasciando senza questo strumento il 21,3 per cento della popolazione italiana, dunque quasi 13 milioni di esseri umani, soprattutto nel Mezzogiorno. Certo, ci sono poi anche biblioteche di eccellenza che hanno a disposizione oltre 10.000 volumi, ma le librerie sono

soggetto a rincari che avrebbero messo i librai in una condizione di inferiorità rispetto alla grande distribuzione. In quell'occasione fu dunque

suggerito con riferimento al testo mutuato dalla Camera dei deputati. Tra l'altro, a dimostrazione che mettere un tetto, ancorché molto definito e non esagerato, è importante, valga l'esempio al contrario del Regno Unito e dell'Irlanda, in cui una a nostro modo di vedere - dissennata liberalizzazione selvaggia non ha portato ad un aumento del consumo culturale, ma anzi ad una riduzione netta del numero delle lettrici e dei lettori.

un doveroso compromesso tra una politica pubblica ed un giusto e doveroso riconoscimento al mercato e del mercato. Altrettanto si può dire del tetto alle vendite promozionali,

o di statalismo. Al contrario, è un modo per favorire quella parte di mercato che non ha le stesse regole delle merci qualsiasi, in quanto attiene alla nostra coscienza più profonda, all'essere cittadini. Se si è più colti, si è più cittadini. Se si legge di più, finalmente l'Italia avrà un peso maggiore di quello che dice il suo PIL.

ciò è fondamentale. Chi non l'ha regolamentato, come ad esempio l'Inghilterra, oggi ne paga le conseguenze, ed anche amaramente. Detto questo, entro nel merito

anche se tale disposizione ha avuto un *iter* assai accidentato. La relativa entrata in vigore è stata infatti più volte rimandata con una serie di decreti-legge, fino a quando nel 2006 non è rientrata nelle liberalizzazioni promosse dall'allora ministro dello sviluppo economico Bersani. La cancellazione di tutti i vincoli della distribuzione commerciale per le attività di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 ha incluso infatti anche il settore dei libri. per tale comparto sono stati aboliti i limiti riferiti alle vendite promozionali e alle connesse autorizzazioni preventive, tanto che il settore ne risulta fortemente deregolamentato. Ecco il motivo per il quale nasce questo disegno di legge, richiesto da tutti. Come si è detto, tuttavia, la totale liberalizzazione del settore in altri Paesi - lo ricordo - come il Regno Unito, ha dato esiti negativi, provocando una impennata dei prezzi e la chiusura delle piccole librerie. Vorrei ricordare la figura del librario, che spesso dimentichiamo. È un uomo di cultura che, prima di noi, legge i libri e si informa sui testi. Chi desidera

Ecco la motivazione vera dell'equilibrio tra grandi editori, piccoli editori, grande distribuzione e piccola distribuzione, cioè il libraio.

reintroducendo nell'ordinamento una normativa assai simile a quella a suo tempo recata all'articolo 11 della legge n. 62 del 2001. In particolare, si è cercata una via mediana, che componesse gli interessi degli editori più grandi, da sempre favorevoli ad un prezzo di vendita totalmente libero, e quelli degli editori più piccoli e indipendenti, che propendono per un prezzo fisso senza possibilità di sconti. disegno di legge arriva ad un equilibrio tra queste due esigenze estreme. L'originaria proposta dell'onorevole Levi della Camera dei deputati prevedeva perciò la fissazione di un tetto massimo agli sconti, pari al 15 nonché la possibilità di sconti ulteriori nel corso di campagne promozionali, la cui durata massima era fissata in un mese. In questo modo, si forniva una cornice più definita nell'ambito della quale poter svolgere attività di promozione del libro e della lettura. A seguito degli emendamenti approvati dalla Commissione cultura dell'altro ramo del Parlamento, tuttavia, l'opportunità di svolgere campagne promozionali è stata estesa undici mesi all'anno, con la sola esclusione del mese di dicembre. L'altra novità del provvedimento licenziato dalla Camera dei deputati rispetto al testo del 2001 riguardava l'editoria scolastica, che risultava inclusa nell'applicazione della legge.

Assai opportunamente sono stati infatti auditi i rappresentanti dei diversi soggetti interessati dalla legge, sia i grandi sia i piccoli editori, nonché i librai, ivi inclusi quelli indipendenti. Le posizioni emerse sono apparse diversificate, ma non inconciliabili. Ad esempio, si è registrata un'ampia disponibilità alla fissazione di un tetto anche per gli sconti ulteriori, nonché ad una migliore definizione delle promozioni. È altresì emersa la comune preoccupazione per la crescente fetta di mercato raggiunta dalla grande distribuzione, in particolare dai supermercati, dove sono possibili sconti tali da snaturare le caratteristiche proprie del libro. riscontrava il più ampio e trasversale consenso sulla predetta linea e accoglieva dunque, nello scorso mese di novembre, alcune modifiche al testo già licenziato dalla Camera dei deputati, richiedendo alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante. Va segnalato peraltro che era stato introdotto anche un inasprimento delle sanzioni. Successivamente, tuttavia, emergevano alcune difficoltà, specificamente connesse al conseguimento del prescritto assenso del Governo per il trasferimento di sede. Fra l'altro, si manifestava l'esigenza di una modifica della disciplina delle vendite per corrispondenza, ancorché effettuate *on line*. I due correlatori si sono così adoperati in un'intensa attività di mediazione per superare l'*impasse* che si era determinata e giungere ad una sollecita approvazione della legge, largamente attesa dagli operatori di settore. In particolare, sono stati svolti numerosi incontri, anche con i rappresentanti dell'Esecutivo nonché delle case editrici e dei librai, per trovare una soluzione soddisfacente rispetto a tutte le esigenze in campo, che al contempo fosse condivisa dall'altro ramo del Parlamento, al quale - occorre rammentare - spetterà la terza lettura del disegno di legge. Non va dimenticato peraltro che, nelle more di conseguire il consenso del Governo al trasferimento alla sede deliberante, la Commissione aveva anche prospettato la possibilità di portare il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, onde velocizzarne l'*iter*, ottenendo tuttavia un diniego. Nel frattempo, interveniva a metà novembre la sessione di bilancio, che impediva la trattazione di qualunque provvedimento comportante spesa e imponendo perciò una forzosa battuta d'arresto. Il testo contiene infatti un articolo 4 secondo cui i comuni provvedono alle attività di vigilanza che competono loro, nonché all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle eventuali sanzioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la cui neutralità finanziaria deve essere certificata dalla 5a Commissione permanente. Com'è noto, dopo l'approvazione della legge di stabilità il Parlamento è stato impegnato, a metà dicembre, con la verifica della fiducia al Governo in carica indi, il Senato si è dedicato all'approvazione della legge di riforma universitaria. L'*iter* del disegno di legge sul libro è rimasto quindi purtroppo fermo fino alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa natalizia. E stato perciò con viva soddisfazione che, nella seduta del 15 febbraio 2011, i due correlatori hanno potuto annunciare alla Commissione di aver raggiunto un'ampia intesa su alcuni ulteriori ritocchi da apportare al testo, tali da consentire di ottenere l'assenso del Governo alla sede deliberante ed una celere approvazione anche presso l'altro ramo del Parlamento. In particolare, si suggeriva di applicare lo sconto massimo del 15 per cento anche alle vendite di libri per corrispondenza, quelle cosiddette *on line*, Inoltre, con riguardo alle campagne promozionali, si proponeva di ridurre ad un quarto del prezzo fissato la percentuale massima di sconto, mentre precedentemente, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, per le promozioni non era fissato alcun tetto allo sconto e si poteva quindi raggiungere anche il 90 impossibile per i piccoli librai e i piccoli editori raggiungere quella cifra. Quanto all'entrata in vigore, considerati i tempi presumibili di approvazione definitiva, si suggeriva di posticiparla al 1° settembre 2011. Ritenendo essenziale monitorare l'applicazione della nuova disciplina, tra le modifiche si prevedeva altresì un'indagine conoscitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i cui risultati sarebbero stati comunicati al Parlamento. Infine, si segnalava l'esigenza di ritornare alla stesura precedente con riguardo alle sanzioni e all'editoria scolastica, onde corrispondere ad alcune perplessità da più parti manifestate. Di questa intesa veniva debitamente informata la Presidenza del Senato, affinché la rappresentasse formalmente al Governo ai fini dell'espressione del consenso alla sede deliberante. Il provvedimento è stato invece calendarizzato dalla Conferenza dei rappresentanti dei Gruppi in Assemblea. I due correlatori I due correlatori si sono pertanto fatti carico di presentare alcuni emendamenti che riproducono l'intesa sopra descritta e di cui raccomandano perciò vivamente l'approvazione da parte dell'Assemblea. Nel manifestare qualche rammarico per la mancata conclusione dell'*iter* in Commissione, tanto più alla luce del consenso unanime manifestato sul punto da tutte le forze politiche, come recentemente rilevato anche dal senatore Giambrone in Commissione, nonché dell'imminente compimento di tutti i passaggi procedurali, i correlatori si compiacciono comunque che il provvedimento giunga alla fase di approvazione, esprimendo l'auspicio che l'altro ramo del Parlamento possa sollecitamente licenziarlo in via definitiva. Il settore avrebbe così finalmente una legge largamente attesa, in un testo final-mente ampiamente condiviso, a riprova di come il legislatore sappia ben lavorare su temi di interesse comune, con la proficua collaborazione di tutte le forze politiche.

*(PD)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, relatori, la storia del libro e l'importanza che ha avuto per la nostra cultura sono state ampiamente illustrate illustrate nelle due relazioni che abbiamo testé ascoltato. Voglio affrontare la questione che secondo me è più rilevante. Sono preoccupato per l'assenza del Ministero dei beni culturali a questo dibattito, seppur breve, su un tema così importante, perché la vicenda è più rilevante di quello che appare. Ho avuto dubbi rispetto al testo, perché si tratta di un testo che va ad indicare limiti massimi nella scontistica

una limitazione alla libertà economica ed alla competizione, a quella che considero una sana dialettica tra la domanda e l'offerta, in un settore merceologico che però ha caratteristiche specifiche rilevanti, che è opportuno sottolineare:

debbano mettere in parallelo le considerazioni sulla libertà economica rispetto alla libertà di espressione e culturale e al valore che queste hanno all'interno di un quadro generale valoriale di un Paese.

si ha una spiccata, indefinita, non regolamentata competizione sul prezzo del libro, in realtà, dopo pochi anni di *dumping* all'interno delle librerie e di una competizione tendente non a dare al minor prezzo possibile il miglior prodotto possibile all'utente finale, a comprimere il numero dei *competitor* nel settore, si è creato un meccanismo di oligopolio spinto, che ha portato non all'abbassamento dei prezzi dei libri e quindi alla facilitazione della loro divulgazione nella

a supporto di tutti i cittadini, in particolare nei centri di provincia e nei luoghi dove non esistono le grandi librerie. librerie. Vi è un meccanismo culturale che si andrebbe a limitare, o forse ad incrinare definitivamente, se si permettesse alle grandi case editrici e alle grandi catene di librerie di librerie di considerare questo settore merceologico come uno qualsiasi, che è indipendente dagli altri fattori e che non ha un valore aggiunto rispetto alla qualità della vita percepita all'interno di un Paese. Credo che la dialettica che vi è stata tra i due rami del Parlamento e all'interno della Commissione, tra maggioranza e opposizione e con lo stesso Governo sia stata proficua: ha tenuto conto delle esigenze complessive della società ed anche delle esigenze di settori diversi, forse i più deboli della cultura di questo Paese. Mi riferisco alle culture territorialmente limitate che trovano espressione nelle piccole case editrici, ai giovani autori che altrimenti non troverebbero un editore che provveda alla edizione dei propri libri, libri, a situazioni diverse che altrimenti sarebbero indebolite. Sarebbe facile, forse, per l'autore affermato avere una maggior distribuzione e forse maggior utenza e vendite, e sarebbe sicuramente molto più problematico per i più deboli avere accesso alla edizione. Queste ragioni mi portano a pensare che quello in esame sia un buon provvedimento. Non si raggiunge un un effetto secondario ma un effetto principale: quello di tutelare il pluralismo culturale, di tutelare le piccole case editrici, di tutelare gli autori che in numero sempre maggiore - mi auguro - possono avere pubblicati i loro libri, di tutelare le piccole librerie e le comunità più deboli. Credo che in questa logica si possa confluire anche nel sacrificio - lo sottoscrivo come sacrificio di limitare la libertà economica degli operatori del settore, di non permettere un'aggregazione troppo spinta e comunque di tutelare secondo me un valore aggiunto complessivo per la nostra società. Non ci possiamo dimenticare che ormai dimenticare che ormai siamo da alcuni anni in una realtà diversa, dove vi sono fonti diverse di distribuzione della cultura, e nello specifico Credo che questo provvedimento, una volta approvato nel testo che propone la Commissione con gli emendamenti previsti e sottoposti all'attenzione dell'Aula da parte dei relatori, dei relatori, ci permetterà di avvicinarci a quel mondo in maniera graduale, mantenendo il maggior numero di attori vivi in un settore culturale ahimè messo alla prova troppo duramente in questi anni: è stato troppo penalizzato dalla politica di questo Governo. Quindi, da parte mia vi è un contributo, un supporto al lavoro svolto da parte dei relatori, un apprezzamento per quello che è stato fatto e una favorevole sul provvedimento in esame, che va a salvaguardare quello che è ancora possibile salvaguardare in questo difficile settore culturale per il nostro Paese.

in modo particolare il Comune di Casette d'Ete e le province di Fermo e Ascoli Piceno. Ci sono stati, a questo momento, tre morti per l'esondazione del fiume Ete. Un evento meteorologico di intensità forte sta mettendo in ginocchio un territorio importantissimo per l'economia, in questo momento molto fragile, della nostra Regione. Chiedo quindi a tutti - a lei, Presidente, e

intervengo relativamente all'informativa che questo pomeriggio il ministro La Russa renderà circa gli ultimi accadimenti in Afghanistan (è già accaduto in occasione dell'informativa del ministro Frattini). Ritengo, proprio perché siamo reduci da un dibattito sul pluralismo culturale, che attribuire cinque minuti per Gruppo per rispondere a qualcosa che sarà sì e no sì e no una rielaborazione di fatti arcinoti non sia all'altezza dei problemi che invece saranno al centro della relazione del Ministro stesso. Abbiamo potuto apprezzare la flessibilità della Presidenza la settimana scorsa. Credo che sarebbe opportuno poterla apprezzare di nuovo in questa circostanza, che, durante il dibattito relativo alla proroga delle missioni internazionali, è stato fatto proprio da parte del Governo un ordine del giorno in cui ci si impegna ad affrontare il prosieguo del dibattito circa la presenza italiana all'estero in un contesto normativo in cui si arriva a valutare nel merito le missioni internazionali. Oggi espelliamo sistematicamente la possibilità di avere un dibattito e reincludiamo delle informative all'interno dei nostri lavori. Visto che i nostri lavori

nuova finestra"). Sicuramente la Presidenza, come è già avvenuto sull'informativa Libia, avrà un atteggiamento sensibile, stante l'importanza del dibattito.

le gravi irregolarità che sarebbero emerse durante le elezioni amministrative svoltesi a giugno 2009 nel Comune di Gragnano, in provincia di Napoli. Dalle inchieste in corso sarebbero emersi non solo, con grande evidenza, la presenza di voto di scambio, ma anche il sospetto che ci siano infiltrazioni che ci siano infiltrazioni camorristiche. D'altra parte, quest'inchiesta è fortemente intrecciata con l'altra importante inchiesta che si sta svolgendo nel Comune di Castellammare, dopo l'omicidio di un consigliere comunale. Anche quell'inchiesta sta portando alla luce fatti particolarmente inquietanti. L'inchiesta di Gragnano sta andando avanti, ci sono molti interrogatori. Nel frattempo la magistratura ha preso una decisione rispetto alla posizione del Presidente del Consiglio comunale di quella

faccia chiarezza dal punto di vista della politica su questa vicenda, senza interferire, naturalmente, con l'inchiesta che giustamente sta andando avanti e deve andare avanti. Penso però che i cittadini di Gragnano e della provincia di Napoli debbano essere messi a conoscenza anche dalla politica delle cose che lì non sono andate o non vanno. Presidente, anche a nome dei colleghi Antezza e Chiurazzi, chiedo al Governo di riferire in Aula sui provvedimenti che intende adottare o sta adottando in relazione alle situazioni di eccezionale avversità atmosferica che si sono determinate a seguito delle piogge

determinato l'isolamento della Regione Basilicata per effetto dei danni che si sono determinati, su importanti arterie stradali e ferroviarie. La Basentana, l'unica arteria che collega la Regione Basilicata alla rete viaria nazionale, è interrotta per effetto del cedimento di numerosi piloni che consentono appunto il collegamento con il resto del Paese. La ferrovia nel tronco Taranto-Crotone risulta interrotta nell'area metapontina, e nel tratto Taranto-Napoli risulta bloccata in relazione all'area interessata dalla Basentana. La città di Matera è isolata sul versante Potenza e sul versante Puglia; il patrimonio dell'UNESCO risulta messo in una situazione di pericolosità, e migliaia di ettari nel Metapontino risultano invasi dall'acqua; in alcuni punti vi sono addirittura tre metri d'acqua. In dodici ore, signora Presidente, in quella Regione è caduta una quantità di pioggia che è pari al 70 per cento della piovosità media annuale. Questo ha creato problemi: sono crollati ponti sulla viabilità provinciale, isolando Comuni come Montescaglioso, Montalbano, Grassano, Ferrandina, Pisticci, Marconia, l'area del Rionerese e la parte della Val d'Agri. In buona sostanza, siamo di fronte a una situazione di grave difficoltà che viene efficacemente fronteggiata dalle strutture della Protezione civile regionale e dalle amministrazioni provinciali, le quali, però, non avendo le risorse per garantire la gestione ordinaria della rete viaria, oggi vivono questo ulteriore disagio dovendo garantire la circolazione e l'accessibilità per intere comunità. Per questo vorrei pregarla di chiedere al Governo di riferire in Aula in una delle prossime sedute sui provvedimenti che si intende adottare.

per ciò che è accaduto in questa Regione, in particolare nella vallata dell'Ete, che peraltro non è nuova agli sconvolgimenti dovuti al clima e alle intemperie che si abbattono ciclicamente su questo territorio. La situazione, che è stata già in qualche modo riferita dall'intervento, pur breve, del senatore Casoli, è in effetti molto più complessa, perché riguarda una realtà che, dal punto di vista idrogeologico, non è assolutamente attrezzata a sopportare questi eventi climatici così improvvisi

Sappiamo con certezza che la Protezione civile delle Marche è dotata di un'ottima struttura organizzativa ed è efficiente sul piano dell'immediata capacità di approntare tutte le sue risorse per affrontare queste situazioni. sappiamo anche che il responsabile regionale, dottor Roberto Oreficini, ha chiesto lo stato di emergenza. Noi vogliamo dire qualcosa di più: probabilmente non basterà neanche questo, occorrerà dichiarare lo stato di calamità. Chiediamo inoltre che il Governo venga a riferire in quest'Aula, tramite il Ministro dell'ambiente, sulle politiche non solo emergenziali ma di medio e lungo periodo - quindi quelle che hanno degli obiettivi di fronte ai cambiamenti climatici ai quali stiamo assistendo e che sconvolgono le nostre realtà dal punto di vista geografico e orografico - e sulle iniziative che il Governo intende adottare per affrontare queste emergenze dovute al cambiamento climatico che si abbattono soprattutto su Regioni che, ripeto, già strutturalmente hanno rivelato una fragilità nei confronti di questi eventi.

Anche a lei, senatrice Sbarbati, rispondo che la prossima Conferenza dei Capigruppo, convocata su sollecitazione dei vari Gruppi, mi pare la sede più opportuna per calendarizzare non solo un'informativa ma probabilmente anche un dibattito

in relazione anche alle finanze degli enti locali e in particolare dei Comuni. Spero che il Governo possa direttamente valutare gli interventi più congrui per scongiurare che